contiene un intervento ampio e articolato sulle nostre Forze di polizia, sulle Forze armate e sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta di misure che rispondono a necessità di modernizzazione, di ottimizzazione delle risorse e di miglioramento della funzionalità di questi corpi, i quali incarnano il pilastro della sicurezza e della protezione dei cittadini. L'obiettivo del provvedimento è rafforzare l'efficacia organizzativa e operativa di queste istituzioni, introducendo novità che toccano ambiti essenziali: dall'organizzazione interna e i criteri di assegnazione, fino alla semplificazione delle procedure di formazione e reclutamento. In una fase storica in cui l'Italia affronta sfide complesse e il sistema di sicurezza è messo alla prova, è indispensabile un quadro normativo chiaro e aggiornato che permetta a queste Forze di rispondere con prontezza e adattabilità. Con questo intervento, inoltre, si pone un'attenzione particolare ai diritti e al benessere del personale e delle loro famiglie. Dalla possibilità per gli psicologi di svolgere attività libero-professionale all'assistenza per i familiari di agenti caduti in servizio, emerge la consapevolezza di quanto sia essenziale tutelare chi quotidianamente tutela noi. altresì di semplificare l'organizzazione riducendo i tempi di formazione e aggiornando i requisiti di servizio e di trasferimento. Per quanto riguarda le disposizioni rientranti nell'ambito di interesse della Commissione affari costituzionali, leggerò ora gli articoli che fanno appunto riferimento a tale Commissione. L'articolo 1 modifica l'ordinamento della Polizia di Stato. Stabilisce un servizio minimo di quattro anni (due in sedi disagiate) per agenti e funzionari appena assegnati e autorizza incarichi dirigenziali in deroga per cinque anni. Durante il Giubileo 2025 si elimina il requisito minimo di permanenza per i trasferimenti. L'articolo 2 definisce i requisiti per l'accesso ai gruppi sportivi della Polizia e autorizza il reclutamento di familiari di agenti deceduti o inabili. L'articolo 3 permette agli psicologi della Polizia di esercitare la libera professione senza vincoli di incompatibilità. L'articolo 4 riduce i tempi dei corsi di formazione per il personale della Polizia, con estensione del tirocinio per alcune qualifiche. L'articolo 7 modifica l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, stabilendo nuovi criteri per promozioni e graduatorie. L'articolo 8 adegua l'organizzazione della Polizia penitenziaria, precisando le norme su impieghi specifici di personale maschile e femminile. L'articolo 12 concede al Governo una delega per il riordino del Corpo dei vigili del fuoco, senza nuovi costi pubblici, per ottimizzare funzioni e ruoli. L'articolo 13 specifica il diploma necessario per l'accesso ai ruoli del Corpo dei vigili del fuoco entro la data della prima prova. L'articolo 14 autorizza 54 nuove assunzioni nei Vigili del fuoco tramite graduatorie interne e, durante il Giubileo 2025, sospende il requisito di permanenza in sede per i trasferimenti. L'articolo 16, che trasforma il Fondo di assistenza della Polizia di Stato in una fondazione privata, adesso sarà soppresso con un emendamento appunto soppressivo di tale articolo. L'articolo 17 istituisce la Giornata nazionale delle vittime del dovere, con iniziative commemorative, inclusi incontri scolastici per rafforzare l'identità nazionale, senza nuovi costi pubblici. Lascio la parola al collega Dreosto per gli articoli di competenza della sua Commissione.

Signora Presidente, come è stato detto, come relatore della 3a Commissione mi limiterò all'illustrazione dei contenuti di cui agli articoli 5, 6, 9, 10, 11, 15, 18 e 19, che recano profili di interesse per il comparto della Difesa. In particolare, nell'ambito del Capo I, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 5 dispone l'accorpamento in un'unica posizione, quella del Comando unità mobili e specializzate dell'Arma dei carabinieri, retta da un unico generale di corpo d'armata, delle due posizioni di vertice precedenti, il Comando unità mobili e il Comando unità specializzate, che secondo la normativa vigente - erano dirette appunto da due distinti generali di corpo d'armata. Questo al fine di recuperare una posizione di impiego di un generale di corpo d'armata, che sarà poi destinato all'incarico di *manager privacy*, figura che assicura il rispetto e l'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati personali nei processi sviluppati da tutte le unità organizzative dell'Arma dei carabinieri. Per quanto riguarda il comma 2, il medesimo articolo dispone poi che il vertice del comparto contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei carabinieri possa essere, oltre che un generale di brigata, anche un generale di divisione. Il successivo comma 3 dell'articolo 5 consente di far affluire, sul conto corrente fruttifero acceso presso Cassa depositi e prestiti, le somme annualmente maturate a titolo di IVA a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, che sono già affidate al Corpo forestale dello Stato, ora attribuite invece all'Arma dei carabinieri. Da ultimo, il comma 4 dell'articolo 5 interviene sul Fondo per le esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati. sequestrati. L'articolo 6 reca disposizioni in materia di personale del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, finalizzate ad incrementare di 40 unità il personale stesso del Comando. Sempre nell'ambito del Capo I l'articolo 9, che era già articolo 4, contiene diverse norme in materia di personale delle Forze armate, relative in particolare al computo dei periodi dei comandi degli ufficiali in incarichi qualificanti presso enti ed agenzie esterne della Difesa e alla decorrenza delle promozioni a tenente colonnello. Viene introdotta poi dall'articolo 10 una disposizione in materia di personale dell'Arma dei carabinieri, finalizzata ad autorizzare l'Arma all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato in misura non superiore alle 100 unità per l'anno 2025 e alle 38 unità per l'anno 2026. L'articolo 11, introdotto anch'esso con l'approvazione di uno specifico emendamento nelle Commissioni riunite, reca disposizioni in materia di trattamento economico in favore del personale del comparto difesa e sicurezza, finalizzato ad estendere l'incentivo delle funzioni tecniche anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali. È riportato tutto nello specifico allegato. L'articolo 15 reca disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto e della Guardia costiera, prevedendo, a questo fine, di potenziare l'apporto di competenze e di destinare ulteriori unità di proprio personale in questo ambito. Concludo con gli articoli 18 e 19. L'articolo 18 reca alcune modifiche normative dedicate al tema dell'utilizzo delle economie di gara, che possono essere riutilizzate, mentre l'articolo 19 reca alcune modifiche alle disposizioni sulla disciplina degli enti circoli della Marina militare.

devo dire che questo provvedimento era stato accolto dal Gruppo con favore in Commissione. Anzi, direi di più: abbiamo anche cercato di dare un contributo costruttivo di idee per migliorarlo. Però non possiamo non esprimere il nostro rammarico per il fatto che siano stati respinti tutti i nostri emendamenti: un

nettamente contrapposta. In quel caso lo posso capire. Ma, quando siamo in sintonia, che senso ha una tale presa di posizione che va a calpestare i diritti delle opposizioni?

di un'anticipazione del presidenzialismo? Forse è questo, Presidente, perché altrimenti non si comprende per quali ragioni, in un tema in cui pressoché tutte le forze politiche sono d'accordo, voi non date alcuno spazio di miglioramento alle forze di opposizione. Le Forze di polizia, le Forze armate e i Vigili del fuoco si sono fatti carico di una grande responsabilità, perché sono loro che si devono occupare del rispetto delle leggi e della nostra sicurezza. però, Presidente, non deve diventare un pretesto per il Governo per occuparsi di quei problemi sociali e di quel contesto socioeconomico che spesso è la causa da cui originano tali problemi. Il Governo sembra dimenticare che le condizioni di disagio e di povertà sono terreno fertile per la nascita di quella microcriminalità di sopravvivenza e, se non si interviene sulle cause dei problemi, non si può delegare tutto semplicemente alle Forze dell'ordine. State seguendo una politica del manganello, quella repressiva. Non vi occupate dei problemi della gente che non ha casa, non vi occupate della crisi abitativa. Vi preoccupate semplicemente di creare sanzioni più forti per quelli che occupano una casa per non vivere in strada. Dite di voler garantire la sicurezza e demandate giustamente alle Forze dell'ordine. Ma non vi preoccupate, ad esempio, di ridurre il tasso di recidiva in carcere ed è così che persone che non vengono rieducate tornano in libertà e continueranno a delinquere. È questa la sicurezza che volete? Come pensate di rieducare persone che protestano in carcere perché c'è un sovraffollamento sovraffollamento carcerario che non consente il reinserimento sociale e la rieducazione? Come pensate di garantire la sicurezza se non si interviene su quello, e si interviene semplicemente per reprimere anche le proteste pacifiche di chi si rifiuta di entrare in una cella, perché ci sono già altri otto detenuti e in nove in piedi non si riesce a stare? Presidente, tramite non c'è chiarezza di cosa significhi garantire la sicurezza. Noi sicuramente siamo favorevoli a questo provvedimento. Non siamo favorevoli alle politiche complessive del Governo, che sembra

Voi pensate che il cittadino sia più sicuro perché magari un ladro starà un po' di tempo in più in carcere. Ecco, quel cittadino si sentirà molto più sicuro se nello Stato italiano nessuno dovrà più avere bisogno di andare a rubare in un appartamento, perché lo Stato si occupa anche degli aspetti socioeconomici.

dare sicurezza agli italiani, c'è bisogno di un Governo che garantisca un sistema sociale funzionale; che garantisca che non ci siano 6 milioni di poveri e non faccia finta invece che non esistono.

rispetta il dialogo democratico e le opposizioni. Sappiate che, dietro alle opposizioni, c'è una fetta molto importante della popolazione. E, se voi sbattete la porta in faccia a noi dell'opposizione, state chiudendo la porta in faccia a quella popolazione che noi cerchiamo di rappresentare.

quotidianamente, dovete intervenire in quelle sacche di disagio sociale, dove la povertà è una delle principali cause della criminalità. Se non intervenite lì, tutto il resto è fatto soltanto di parole.

occasione di parlare di un tema abbastanza complicato, piuttosto articolato e molto tecnico come quello che è contenuto nel provvedimento È chiaro che con questo intervento vogliamo dare anche un particolare riconoscimento e ancora oggi vogliamo ribadire un ringraziamento a tutte le Forze dell'ordine per quello che stanno facendo nel nostro Paese, dai singoli atti quotidiani alle grandi operazioni. E, quindi, adottiamo un provvedimento, quello di oggi, che è volto sostanzialmente a un migliore efficientamento e a una migliore organizzazione dell'attività interna del complesso sistema dell'ordinamento delle Forze dell'ordine. È difficile, per certi versi, su su questo testo poter fare della politica anche spicciola. Emendamenti su questo provvedimento non sono stati accolti: si tratta comunque di un provvedimento di un altissimo livello di tecnicismo. Non possiamo, però,

il comparto della sicurezza è stato lasciato a sé stesso per trovarsi poi con problemi dai più semplici, come possono essere quelli degli organici, per arrivare anche a quelli più complessi all'interno dello stesso sistema. Anche semplicemente prevedere per la Polizia di Stato che il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione sia di quattro anni invece che di due anni crea un particolare efficientamento all'interno del sistema,

che egli stesso ha fatto. Vi sono poi delle altre previsioni veramente molto importanti per quanto riguarda anche l'Arma dei Carabinieri.

ma anche di quella che può sembrare una questione periferica rispetto all'importanza di altri temi, che è l'accoglienza degli animali sequestrati e confiscati dal Comando unità forestali.

l'appassionato che magari fino a ieri avrebbe voluto custodire o allevare animali

al fine di evitare che vi siano delle norme fini a sé stesse, che si chiudono in sé stesse, senza tener conto di quello che può essere il processo. Anche in questo caso dobbiamo solo ringraziare il Governo per aver finalmente rivolto una particolare attenzione

così complesse e per certi versi anche incomprensibili, forse anche alla stessa magistratura. Abbiamo visto finalmente un Governo che prende anche posizione.

il poliziotto o il carabiniere che si ritrova contuso, aggredito o leso non è lì per creare la rissa, ma è lì per proteggere

modificando in gran parte normative anche vetuste, a dimostrazione del fatto che il Governo è dalla parte delle Forze dell'ordine. Al di là di quanto dice qualche esponente dell'opposizione, per cui vi è solo una politica del manganello, c'è una politica che, dopo tanti anni, ha migliorato i contratti di lavoro delle Forze di polizia: sono migliorie degne di questo nome, perché contratti così non se ne vedevano da anni.

- di stabilire dei punti per ognuna delle Forze dell'ordine, delle Forze di polizia e militari che vengono coinvolte nel provvedimento. Comincio dalla Polizia di Stato, laddove si prevede che l'istituto superiore diventi una scuola, retta da un prefetto, un dirigente generale.

sulle destinazioni dei poliziotti per garantire la sicurezza della città eterna. Sul reclutamento, questo è un provvedimento che guarda con riconoscenza alle Forze dell'ordine, anche

per una forma di riconoscenza a chi ha dato la vita per servire lo Stato. Sulla riduzione dei corsi di formazione, ci sono scuole di pensiero diverse, ma la riduzione del tempo dei corsi di formazione ha il solo ha il solo obiettivo di avere subito i poliziotti in strada. D'altra parte, i cittadini ci chiedono sicurezza e in questo modo si garantisce comunque la formazione ottimale dei nuovi agenti, potranno essere messi subito in servizio e assegnati soprattutto nelle località dove c'è maggiore richiesta di sicurezza. Per chiudere, sulla Polizia di Stato, un aspetto sociale di questo provvedimento è che il Fondo di assistenza diventa una fondazione di diritto privato, che garantirà assistenza scolastica agli orfani e sovvenzioni per malattia ai ai congiunti dei poliziotti che hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere. Tutti i Corpi vengono toccati dal provvedimento. Anche per l'Arma dei Carabinieri intervengono sostanziali modifiche, intanto in generale sulla normativa di categoria. Ma spicca una norma che prevede l'adeguamento, anzi un aumento di contingente speciale per i Carabinieri per la tutela del patrimonio, a dimostrazione del fatto mira alla sicurezza *tout-court*, e per sicurezza intendiamo anche la tutela del nostro straordinario patrimonio artistico. Sulla Guardia di finanza, oltre alle norme strutturali, si incide si incide sulle promozioni, in modo tale da escludere fattori esogeni che possano impattare negativamente sulla promozione degli ufficiali e, quindi, per garantire un'imparziale progressione di carriera. Polizia penitenziaria, anche qui andiamo a modificare una norma che ha oltre trent'anni di vita e dobbiamo dire che, dopo aver stabilito con la finanziaria del 2023 l'assunzione di mille nuovi agenti per garantire la sicurezza nelle carceri (anche questo non accadeva da anni), abbiamo stabilito noi - il Governo Meloni ha stabilito - la parità retributiva tra agenti di sesso maschile e femminile. Anche questa è una novità e anche in tale caso ci è voluto un Governo di centrodestra per garantire parità tra uomini e donne. Sui Vigili del fuoco si incide intanto sul reclutamento, stabilendo che è necessario il diploma di scuola superiore già all'atto della prima prova, ancorché preselettiva. Ma si assumono anche 54 nuovi ispettori antincendio per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini italiani.

(New York, Singapore, Panama e Grecia) per aiutare le nostre rappresentanze diplomatiche. È un provvedimento - checché se ne dica dall'altra parte dell'Emiciclo - a garantire e a migliorare le condizioni di funzionamento e di organizzazione dei nostri Corpi di polizia ed è un provvedimento, come ho detto prima, che guarda anche al senso etico.

consentirà momenti di riflessione e anche di studio scolastico per consolidare il ricordo di chi ha perso la vita in adempimento del proprio dovere. dovere. È un dovere dello Stato, già nelle istituzioni scolastiche, ricordare chi ha servito lo Stato fino all'estremo sacrificio. *(Applausi)*. Ecco perché il Gruppo Fratelli d'Italia non può che guardare con atteggiamento

oggi discutiamo di un tema che tocca il cuore della nostra società, perché la riorganizzazione delle Forze dell'ordine è una questione che riguarda la vita, la dignità e il sacrificio di uomini e donne che quotidianamente indossano una divisa per proteggere tutti noi cittadini. L'efficienza del comparto sicurezza non è solo una questione di risorse, ma anche di strategia e di riorganizzazione che deve funzionare a pieno regime per gran garantire la tutela dell'ordine pubblico, del territorio e dei cittadini. Il principio ispiratore di questo provvedimento può essere sintetizzato così: più flessibilità, più efficienza, più sicurezza. Il disegno di legge che approviamo oggi interviene proprio per rendere più agevole e dinamico il lavoro delle Forze dell'ordine, prevedendo incentivi e meccanismi di collaborazione per fare interagire tutti gli operatori del settore. Interverremo su alcuni aspetti importanti, miglioreremo i benefici assistenziali e snelliremo la burocrazia, semplificando i concorsi per entrare nei vari Corpi dello Stato e rendendo più chiari i criteri per le nomine e le promozioni. Ci teniamo a garantire che gli uffici operativi, che spesso si trovano a fronteggiare carenza di personale, siano coperti in modo efficace. In particolare, sulla gestione delle carriere, andremo a modificare alcune regole sui tempi di permanenza in sede e sulle promozioni, prestando particolare attenzione a chi lavora in zone difficili. Inoltre, per le diverse Forze di polizia, snelliremo i corsi di formazione, riducendo i tempi, pur mantenendo *standard* adeguati. nelle migliori competenze per rendere l'attività investigativa e di *intelligence* ancora più efficace, favorendo uno scambio di informazioni più veloce e flessibile tra le varie Agenzie. Questi sono elementi fondamentali per la prevenzione e la sicurezza dello Stato. Infine, il Ministero della difesa avrà l'opportunità di valorizzare gli ufficiali che si sono distinti per le loro qualità e competenze, permettendo loro di essere impiegati in Agenzie o enti esterni per mettere a frutto le loro professionalità al servizio delle istituzioni, anche in ambito internazionale. Prevediamo inoltre il riordino dell'organizzazione del Corpo dei vigili del fuoco per rendere ancora più efficaci le loro missioni come il soccorso pubblico, la prevenzione degli incendi, gli interventi in caso di calamità naturali, e norme che permettano alle Capitanerie di porto e alla Guardia costiera di rafforzare il controllo e la vigilanza dei nostri litorali. Inoltre, non vogliamo dimenticare i nostri angeli custodi che meritano il nostro omaggio. Ricordiamo sia coloro che hanno perso la vita sia quelli che sono rimasti feriti, così come le famiglie che piangono la perdita di un figlio, di un padre, di una madre, di un fratello, di una sorella. dalle Commissioni riunite l'istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere. Abbiamo anche semplificato le procedure per l'utilizzo dei fondi destinati ad assistere le famiglie degli uomini e delle donne che sono caduti o feriti in servizio. Vogliamo garantire ai loro figli la possibilità di proseguire negli studi e prevedere un sostegno economico in caso di gravi malattie che richiedano cure costose. Oggi approviamo queste norme di buonsenso, frutto dell'ascolto e dei contributi ricevuti dalle associazioni di categoria e dai sindacati delle Forze dell'ordine. Il loro prezioso intervento durante i mesi di discussione al Senato ha permesso di perfezionare ulteriormente questo provvedimento e voglio quindi ringraziarli. Per concludere, questo provvedimento è la dimostrazione più concreta di una maggioranza che crede in chi difende la legalità, valorizza le Forze dell'ordine e le mette nelle condizioni di operare al meglio. Dunque, è questa la differenza tra questa maggioranza e voi dell'opposizione, che oggi forse vi preparate ad una timida astensione, ma fuori da quest'Aula siete quelli che dicono che non è abbastanza. Lo sappiamo anche noi che non è abbastanza, ma per costruire muri servono mattoni e questo è un mattone in più, che mettiamo per creare le condizioni perché lavorino meglio e più in sicurezza, e che andrà ad unirsi alla prossima legge di bilancio. sede verranno stanziati altri 100 milioni di euro per alzare gli stipendi, migliorando la contrattazione e sostenendoli nelle spese legali per i fatti avvenuti in servizio. Voi siete quelli che, mentre una inutile commissione del Consiglio d'Europa accusa le nostre Forze dell'ordine di razzismo, anziché prendere le distanze e stigmatizzare quelle accuse, avete gioito, brindato ed incolpato il Governo, puntato il dito contro chi ogni giorno indossa una divisa dello Stato italiano, si sacrifica e mette tutta la sua passione per garantire la sicurezza di ognuno di noi, in Italia e all'estero. Voi siete quelli che stanno dalla parte degli antagonisti dei centri sociali, che anche in questi giorni, come abbiamo visto a Bologna, vanno in piazza a picchiare i nostri servitori dello Stato; gli stessi manifestanti che scendono in piazza a festeggiare la strage del 7 ottobre da parte di Hamas, aggredendo e lanciando sassi, ferendo esponenti delle Forze dell'ordine diventati bersagli di frustrazioni e violenze che non si meritano. *(Applausi)*. Le abbiamo viste le immagini dei nostri uomini circondati da una folla ostile, costretti a mantenere la calma mentre ricevono sputi e calci negli stinchi, perché non facilmente ripresi dalla telecamera. Anche in questo caso, non abbiamo visto una sola dichiarazione di solidarietà. Voi siete quelli che vogliono smantellare l'esercito in nome del pacifismo solo a parole. Noi, al contrario, vogliamo aumentare la dotazione ed investire nelle Forze armate, perché una Nazione più sicura è anche una Nazione più protetta e pacifica. Per sintetizzare, il vostro modello è Ilaria Salis, picchiatrice di centri sociali, che nel 2023 è stata condannata per resistenza a pubblico ufficiale e per aver insultato e lanciato oggetti contro le Forze dell'ordine. Il nostro modello, invece, è quello della legalità, della sicurezza, della tutela di chi ogni giorno rischia la vita per difendere la nostra. Questi uomini e queste donne non sono solo figure in uniforme, ma padri, madri, figli e amici. Hanno una vita al di fuori del loro lavoro; una vita che spesso viene trascurata a causa delle loro responsabilità. Tutto questo pesa sulle loro spalle, eppure non si tirano indietro mai. La loro determinazione è una testimonianza del loro senso del dovere e dell'amore per il nostro Paese. mio papà ha indossato una divisa per quarantacinque anni, più della metà della sua vita. Oggi compie ottant'anni e quindi dedico questo intervento a lui, che ha avuto come ragione di vita quella di servire il suo Paese.

difesa*. Signora Presidente, prima di entrare nel merito del provvedimento, mi sia consentito oggi, 11 novembre 2024, a sessantatré anni dall'eccidio di Kindu, rendere onore ai 13 aviatori italiani barbaramente uccisi in Congo mentre erano impegnati in una missione di pace nel Paese allora sconvolto dal conflitto dopo l'indipendenza belga. *(Applausi)*. Furono scambiati dai congolesi per mercenari e trascinati dall'aeroporto di Kindu in un piccolo carcere locale, dove il giorno dopo furono barbaramente uccisi. Fu solo un gesto di pietà dell'allora custode del carcere che li seppellì in una fossa comune. Vorrei leggere i nomi di questi caduti: Francesco Paga, Giorgio Gonelli, Giulio Garbati, Filippo Di Giovanni, Nicola Stigliani, Armando Fabi e Antonio Mamone. Vorrei anche ricordare cosa è scritto sul Sacrario di Pisa, che credo sia una frase di altissimo valore: Fraternità ha nome questo Tempio che gli italiani hanno edificato alla memoria dei tredici aviatori caduti in una missione di pace, nell'eccidio di Kindu, Congo 1962. Qui per sempre tornati dinnanzi al chiaro cielo d'Italia, con eterna voce al mondo intero ammoniscono fraternità.

55 milioni di euro stanziati per il trattamento economico accessorio del personale di polizia delle Forze armate. Ricordo anche i 100 milioni di euro stanziati per il pagamento degli straordinari e le norme, con particolare riferimento al Dicastero della difesa e all'Arma dei Carabinieri, per l'assunzione degli operai a tempo indeterminato riferiti al comparto di conservazione e tutela del patrimonio della biodiversità. Va anche annoverata l'assunzione di 40 operatori per la tutela del patrimonio culturale tutte le iniziative volte a rafforzare l'ampia attività dell'Arma dei Carabinieri. Credo sia di altrettanta importanza e valore l'istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere, un sacrosanto

**Il Senato non approva**.

si parla di benefici, di qualsiasi natura, spettanti in base alla vigente normativa alle Vittime del dovere nonché ai familiari; si parla di esenzioni fiscali. Chiedo se non sia da sostenere questo tipo di emendamento, che invito la maggioranza a

Presidente, ancora una volta ci tocca stigmatizzare il ricorso all'articolo 81, perché viene impiegato questo schermo da parte della maggioranza per non assumersi delle responsabilità di merito. La proposta che è stata avanzata, che peraltro ha una dotazione economica risibile dal punto di vista complessivo del bilancio dello Stato - stiamo parlando di 3 milioni di euro - si sarebbe tranquillamente potuta risolvere con un minimo di volontà politica, che evidentemente non c'è stata. Credo che sarebbe giusto che la maggioranza in quest'Aula spiegasse se non c'è stata una volontà politica, perché l'emendamento è stato proposto da un Gruppo dell'opposizione e già questo meriterebbe una stigmatizzazione - o se non si condivide il merito della questione, cosa che sarebbe alquanto preoccupante.

un milione di euro sono veramente un'inezia, dato che abbiamo visto passare disegni di legge d'iniziativa governativa per istituire premi ai cuochi di questo Paese. Con tutto il rispetto, mi chiedo se questa maggioranza, che è così attenta alle nostre abilità culinarie, non abbia la capacità, nelle pieghe del bilancio, di reperire fondi che per altre finalità,

incapacità o all'impossibilità di trovare una copertura finanziaria mi pare che sia veramente poco dignitoso anche per questa Camera. Sentirci dare questo tipo di motivazioni non nobilita il nostro dibattito.

lo dico per i colleghi che non lo hanno letto - tratta di modifiche in tema di contribuzione obbligatoria a carico del personale della Guardia di finanza a favore della Cassa ufficiali del fondo di previdenza, nonché in tema di utilizzo delle economie di gara da parte del Fondo di assistenza stessa. Il Governo esegue

presentato un emendamento che potrebbe benissimo essere il vostro. C'è un fondo di previdenza che, laddove facesse degli utili, servirebbe a comprare titoli di Stato. Non vedo perché dobbiate votare contro un emendamento di questo tipo.

per l'utilizzo di questo fondo, il sentire le organizzazioni sindacali della Guardia di finanza. Questo emendamento semplicemente cambia il consiglio direttivo del fondo, lo porta da cinque a tre membri e dà rappresentanza alla base della Guardia di finanza, togliendo l'ufficiale. Nel momento in cui ci sono da prendere decisioni che riguardano la base della Guardia di finanza, chiedo che ci siano almeno le associazioni sindacali a decidere per il loro futuro. Non dico nient'altro in questo emendamento.

con l'emendamento 19.200 si chiede banalmente che al circolo ufficiali della Marina possano accedere tutti i marinai, indistintamente, senza scegliere tra ufficiali e sottufficiali. Si chiede banalmente questo e che l'iscrizione al circolo ufficiali e sottufficiali non sia d'ufficio, ma sia su domanda dell'interessato.

C'è una sentenza del Consiglio di Stato, che è stata emanata circa un anno fa, che vieterebbe al Ministero della difesa di fare questa sottrazione indebita di parte dello stipendio. stipendio. Nel momento in cui c'è una sentenza del Consiglio di Stato, io mi aspetto che il Ministero della difesa ponga in essere tutto quello che è in suo potere per sanare la situazione.

non vuole partecipare a quei costi, non vedo perché non gli si debba restituire quello che per me è un maltolto. Chiedo quindi al Governo se non sia il caso di porre fine a questa situazione dicendo - come affermato prima ufficiali e sottufficiali hanno il diritto di iscriversi all'ente circolo. Se vogliono, partecipano e pagano la quota; se non vogliono, quella quota non deve essere trattenuta.

qui si chiede banalmente di verificare, al 30 giugno 2025, quello che succede con l'applicazione di questa legge, ossia di fare una relazione al Parlamento per capire quali sono stati i suoi effetti

fra un anno ci ritroviamo e vediamo cosa sta succedendo. Chiediamo una piccola relazione, e non credo costi molto al Governo fare una relazione sull'applicazione di questa legge.

che i giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma hanno sospeso il giudizio sulla convalida del trattenimento dei sette migranti trasbordati sulla nave Libra in Albania, rinviando la questione alla Corte di giustizia europea. Non essendoci dunque, entro le quarantotto ore previste dalla legge, la convalida dei fermi disposti dal questore di Roma, le persone sono libere e, non potendo restare in Albania, come previsto dal protocollo siglato da Giorgia Meloni e da Edi Rama, dovranno tornare in Italia e verranno riportati a Brindisi nelle prossime ore. Signor Presidente, siamo di fronte al secondo *flop* consecutivo di questa vicenda. Mentre noi qui stiamo discutendo, giustamente, di Forze dell'ordine, anche a seguito di questo ennesimo buco nell'acqua, noi abbiamo poliziotti che stanno controllando il nulla in terra di Albania, mentre potrebbero e dovrebbero venire nelle nostre strade, davanti alle nostre scuole, davanti alle nostre stazioni, per svolgere la loro funzione. Di fronte a questa vicenda, noi riteniamo indispensabile che il Ministro dell'interno, anziché insultare i sindaci e attaccare attaccare coloro i quali stanno sul territorio, venga in quest'Aula e ci spieghi che cosa sta realmente accadendo in questo Paese, perché su tale vicenda si sta sfiorando il senso del ridicolo. *(Applausi)*. Chiediamo, pertanto, alla Presidenza di farsi parte attiva affinché su questa vicenda il Governo riferisca immediatamente in Aula. Presidente, anche le galline ormai sanno che i giudici hanno l'obbligo di di disapplicare i provvedimenti che non sono in linea, dal 4 ottobre, con quella sentenza della Corte internazionale di giustizia Ma la furbizia dove sta? La furbizia sta nel continuare a fare questa messa in scena: provocare le sentenze dei giudici, che non possono fare altrimenti, e poi dire che stanno facendo qualcosa e che sono i giudici, cattivi, che non gli permettono di fare quello che vogliono fare. *(Applausi)*. L'astuzia, l'intelligenza malevola: sanno che i giudici sono obbligati e loro fanno questa messa in scena, questa *ammuina*. E la fanno in maniera tale da avere il nemico: che vogliono fare qualcosa, ma i magistrati, cattivoni, non glielo permettono. Guardi, signor Presidente, dove arriva la possibilità di esercitare il potere, ma con i soldi degli italiani! Se questa cosa l'avessero fatta con i soldi loro, noi non avremmo avuto niente da dire. Ma quello in Albania è un centro fuffa per i migranti, per poter dire che si sta facendo qualcosa, dopo che sono entrati 250.000 irregolari in due anni. Le nostre stazioni, le nostre metropolitane, le nostre periferie sono piene degli irregolari entrati in questi due anni di Governo! E non è con l'*ammuina* che riuscite a distrarre l'opinione pubblica. I giudici non c'entrano niente. I giudici stanno facendo il loro lavoro. Siete voi che non state facendo il vostro lavoro!

per sollevare una questione che noi, peraltro, abbiamo sollevato per settimane quando abbiamo trattato il provvedimento sull'istituzione dei centri in Albania. Noi avevamo detto in maniera chiara che cosa sarebbe successo, si sarebbe trasformato in uno *spot* elettorale e nient'altro: solo in uno *spot* elettorale, ma uno *spot* elettorale di 800 milioni. *(Applausi)*. Noi siamo qua a discutere di trovare un milione di euro per le borse di studio per i figli delle vittime del dovere. Stiamo discutendo di tre milioni di esenzioni fiscali per i figli delle persone che hanno perso un proprio caro nell'esercizio delle proprie funzioni. Parliamo di figli di poliziotti e carabinieri.

Ma noi riteniamo la Nigeria un Paese sicuro, senza distinguere da Stato a Stato, quando ci sono gli Stati del Nord che sono in mano a Boko Haram, un'organizzazione terroristica? Come si può pensare di rimandarli in Nigeria, nelle regioni del Nord dove ci sono i terroristi? Come si può pensare che possano ritornare tranquillamente in quel posto? Vuol dire non conoscere la geografia e la storia di quei Paesi. davvero che dobbiate ripensarci, tornare qui e ammettere che questa è una sconfitta che costa ai contribuenti italiani più di 800 milioni di euro e non risolve il problema serio della gestione dei flussi migratori.

che l'Egitto è un Paese sicuro perché un sacco di turisti italiani va a fare le immersioni a Sharm el Sheik. Francamente, cosa si deve aggiungere a questo tipo di considerazioni? *(Applausi)*. Cosa si deve dire oltre a questo?

E magari adesso ci sveglieremo davvero perché…

C'era un famoso *post*, sui *social* del Partito Democratico, che diceva: noi le cose che facevamo le facevamo non nell'interesse degli italiani, ma nell'interesse dell'Unione europea. Certo, lo sappiamo, è sempre stato così: dell'interesse degli italiani non ve ne è mai fregato niente, però per i migranti e per altre cose invece va benissimo. *(Applausi)*. Quindi, è ovvio che adesso un po' se la prendano. Se la prendono perché hanno capito che è stato passato il segno. è stato passato il segno, signor Presidente. Noi qui non possiamo rischiare che ogni legge, se non è gradita a qualche giudice, senza alcun tipo di controllo venga o disapplicata direttamente o rinviata all'Unione europea. *(Applausi)*. Ero rimasto che una volta Ero rimasto che una volta il giudice poteva mandare alla Corte costituzionale. Se io fossi alla Corte costituzionale, proverei vergogna, perché significa che non contano più nulla nemmeno la Consulta; viene scavalcata e si va direttamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La nostra Costituzione non conta più niente

che Paese sicuro potrebbe essere l'Iraq. *(Applausi)*. Eppure sono nell'Unione europea anche a loro. Se il diritto è dell'Unione europea, chi è fuorilegge, noi o loro? Io credo che siano i nostri giudici ad essere fuorilegge. La prossima volta, invece di portarli in Albania, li porteremo a casa di quel giudice, così forse potrà ragionare un po' meglio. Faremo lì il deposito per studiare le cause. State però tranquilli perché, nel caso qualcuno non abbia capito,

però che si è anticipato il dibattito. Pensavo si dovessero fare le dichiarazioni di voto sul provvedimento, ma stiamo facendo un'altra discussione; la cosa mi meraviglia, ma non mi scandalizza, perché il Parlamento è fatto per parlare e quindi chi vuol dire le proprie idee le esprime. Dico quello che avrei detto a fine seduta. Ho assistito in questi giorni, signor Presidente, a numerosi comizi e manifestazioni politiche di magistrati che hanno dato luogo a comizi e manifestazioni politiche, cosa che la magistratura non dovrebbe fare in un mondo normale. *(Applausi)*. al comizio con Santalucia ed altri, che è avvenuto a Bologna giorni fa, a sostegno di non so quale magistrato che aveva emesso un'ordinanza simile a quelle Mi riferisco alla sequela di comizi che abbiamo visto, dal Campidoglio di Roma (nella Sala della Protomoteca) al Congresso sessantennale di Magistratura democratica, preceduto da un magistrale articolo di Facci su «Il Giornale», che manderò a tutti i colleghi senatori. Nel sessantennale della sua costituzione, Magistratura democratica poteva cogliere l'occasione per scusarsi delle dichiarazioni deliranti rilasciate nell'arco di questi sessant'anni, che Facci ha pubblicato su «Il Giornale» e che molti forse non conoscono, di appoggio a qualsiasi situazione di contestazione e di ribellione, dicendo che la magistratura ha il compito questo è lo stillicidio di dichiarazioni di Magistratura democratica - di essere un contropotere, di riscrivere la storia, di opporsi al Parlamento. Ha fatto bene il vice presidente del Consiglio Tajani, poco fa, a dire che la decisione di Roma è un ulteriore atto che contrasta con la tripartizione dei poteri (esecutivo, giudiziario e legislativo). La magistratura ha deciso, in buona parte, di sostituirsi al potere del Parlamento e del Governo, e questa è una scelta eversiva. Uso le parole che vanno usate: è una scelta eversiva. Dopodiché ieri è successa un'altra cosa sconcertante, che volevo dire a fine seduta: la dottoressa Albano, presidente di Magistratura democratica, ieri, intervenendo alla manifestazione politica di MD, in un suo comizio ha anticipato la sentenza di oggi, perché ha detto letteralmente che è stato depositato un verbale. Io l'ho denunciato ieri, senatore Boccia: l'ho detto al telegiornale, l'ho detto in pubblico e lo dico anche il Parlamento, non è un segreto. La dottoressa Albano ha detto che era stato depositato il verbale di una sentenza di un giudice monocratico che avrebbe deciso sulla questione dei sette immigrati. Mi chiedo, e lo dico anche in un'Aula di Parlamento - ho chiesto con un'interrogazione un'ispezione al Ministero della giustizia - come mai la dottoressa Albano sapeva che c'era un deposito di un altro giudice e ha fatto trasparire i contenuti? Era un suo potere? Oppure qui fanno il congresso permanente e si scambiano le carte pure quando scrivono le sentenze che non sono di loro competenza? *(Applausi)*.Siamo di fronte a fatti gravissimi, eversivi dell'ordine democratico e repubblicano, e lo diciamo con nome e cognome! La dottoressa Albano ha accusato Giorgia Meloni di attaccarla. Rispetti il Governo e la democrazia. *(Applausi)*. Qui siamo una Capitol Hill al contrario. La Capitol Hill la stanno facendo i magistrati e qualcuno si metterà anche la pelle di bisonte sulla testa e verrà in Parlamento. Siamo sgomenti per la Repubblica a causa di queste decisioni fotocopia. Il giudice di Bologna, per il quale hanno fatto la manifestazione con Santalucia, ha scritto nella sentenza la famosa frase sulla Germania nazista, secondo cui anche la Germania nazista. L'ha scritto nella sentenza una settimana fa; era la stessa frase che aveva usato un anno prima in una conferenza. Una volta facevano le fotocopie per queste sentenze politiche. Ora con i *computer* fanno il taglia e incolla; ripetono le stesse frasi delle conferenze e trasformano i comizi in sentenze. Questo non si può fare in uno Stato democratico retto da una Costituzione e da principi liberali. Questa è la realtà, cari colleghi. *(Applausi)*. Mi fermo, perché credo che il tempo si sia esaurito, e anche la pazienza. Io credo che in Italia abbiamo bisogno della rifondazione della magistratura, per rendere onore a quei magistrati onesti, le cui inchieste venivano archiviate. *(Applausi)*.Quelli che oggi fanno i satrapi archiviavano le inchieste di Borsellino, che noi riapriremo nella Commissione antimafia,

È successo che un giudice della Repubblica abbia rimesso gli atti alla Corte di giustizia europea, come hanno fatto altri colleghi prima. Non ha disapplicato la legge italiana, ritenendo che la legge europea o meglio una sentenza della Corte della giustizia europea, quella del 4 ottobre, fosse superiore e prevalesse. No, non ha fatto questo. Come altri giudici, ha chiesto alla Corte europea come deve essere interpretato un regolamento dell'Unione europea del 2013 e, cioè, se

Come sappiamo, le sentenze della Corte europea sono vincolanti quanto al dispositivo, non quanto alla motivazione, ovviamente. E il dispositivo della sentenza del 4 ottobre riguarda una fattispecie diversa. È il caso della Transnistria, un Paese nel quale le autorità costituite non hanno il controllo dell'intero territorio perché - come tutti sappiamo la Transnistria è controllata di fatto dalla Russia. Certamente in Transnistria non ci

un Paese o è sicuro per tutti o non lo è per nessuno. Non è vero. Sentiremo cosa dice la Corte europea su questo specifico punto.

Colleghi, capisco tutto, ma dobbiamo anche avere il senso delle proporzioni. La gestione dell'immigrazione, dal gratuito patrocinio all'accoglienza e a tutto il resto, costa all'Italia, guardando il bilancio,

il risparmio che ci consentirà di realizzare la gestione dei migranti in Albania sarà di circa 1,7 miliardi.

Prima che entrasse in vigore il decreto-legge varato dal Governo, i documenti finivano tutti in fondo al mare. È inutile che vi stia a spiegare qual è il vantaggio per un migrante di non rendere noto il Paese da cui proviene, perché chiaramente in questo modo impedisce la procedura accelerata. Non solo, ma c'è stato anche un calo drastico di migranti provenienti dall'elenco dei 19 Stati sicuri, perché chiaramente Internet ce l'hanno anche loro e soprattutto lo leggono non solo i migranti, ma anche gli scafisti che sfruttano e fanno traffico di migranti. Sapete qual è il problema? Noi abbiamo una strategia per limitare l'immigrazione selvaggia e incontrollata e far sì che chi vuol venire in Italia ci venga rispettando le regole e avendo già un lavoro quando arriverà, tant'è vero che sono già migliaia i migranti che vengono formati oggi nei Paesi di provenienza per arrivare in Italia avendo un lavoro, conoscendo l'italiano di questo genere. Voi non avete una risposta, per voi devono venire tutti, cioè 800 milioni di migranti nei prossimi anni. È chiaro che una posizione del genere è insostenibile.

È inutile che ogni volta facciate gli elenchi per dire quali altri Paesi portano i migranti in quali Paesi: non è questo il punto. La Corte europea ha detto che non si può fare un procedimento sommario e accelerato quando si è di fronte a un Paese che non è sicuro in tutte le sue parti e per tutti i gruppi della sua popolazione. un concetto talmente ragionevole che non so come si possa dire che i giudici comunisti applicano questo principio. Si tratta solo di

caso per caso, non è detto che poi il migrante non possa essere riportato anche in quei Paesi. Ha cercato di spiegarvelo il giudice di Bologna

Sarebbe molto semplice: prendete atto del principio che i giudici italiani devono applicare. Il collega Borghi dice che una giudice ha previsto uscita questa sentenza. È chiaro: tutti i giuristi prevedono che escano queste sentenze, e non può essere altrimenti; siete solo voi che non lo capite. Prendetene atto e adeguatevi, invece di lamentarvi dei giudici comunisti e delle toghe rosse, che è completamente fuori luogo.

e il Paese immaginario delle sinistre. Il Paese reale, infatti, la pensa esattamente come noi e voi continuerete a perdere nelle urne, perché non capite che liberare i migranti, che liberare anche anche oggi otto migranti di cui non si sa la provenienza, non si sa se sono delinquenti, terroristi, scappati di casa o scafisti è esattamente quello che gli italiani non vogliono. *(Commenti).* Fate parlare, per cortesia, come vi abbiamo fatto parlare noi: avete fatto un comizio! *(Commenti).* la pensano esattamente come noi. Se non vi rendete conto della delinquenza che viene portata da certa immigrazione e che l'immigrazione clandestina va controllata, continuerete a perdere nel Paese e a farvi difendere soltanto da una parte della magistratura, che non è amata neanche dai magistrati seri di questo Paese.

e soccorso pubblico. Parliamo di interventi in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e di norme in materia di benefici assistenziali in favore del personale del comparto. A una settimana dalle celebrazioni del Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate ci troviamo in quest'Aula per approvare un provvedimento che mira a modificare e attualizzare l'ordinamento di questo settore fondamentale per la vita di ognuno. A loro consentitemi di offrire solidarietà per le violenze e gli attacchi subiti negli ultimi giorni a Bologna (sabato nello specifico) da parte di manifestanti che riconoscono solo a parole della democrazia; finti rivoluzionari che, con il pretesto di sfilare per la pace, scatenano una guerriglia urbana evidentemente preordinata. Sono episodi di una gravità inaudita, da condannare sempre perché commessi contro chi, con professionalità ed equilibrio, è al servizio della Nazione. Sappiamo però che non basta rendere omaggio a chi difende i valori della Patria, baluardo di pace e presidio di libertà e indipendenza, ed esprimere solidarietà se non garantiamo alle donne e agli uomini in divisa un sistema organizzativo moderno, snello e rispondente alle loro necessità ed esigenze di servizio. Senza Forze armate non c'è democrazia, non c'è libertà, non c'è giustizia, né pace. Le sfide di oggi sono complesse e ci impongono un sistema delle Forze che sia in grado di continuare a tutelare l'Italia, soddisfacendo le istanze di chi, con onore e passione, indossa la divisa. Nel dettaglio, per la Polizia di Stato abbiamo nuove disposizioni che regolano il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli agenti in prova, dei vice ispettori e dei commissari di Polizia di Stato: si passa da due a quattro anni in caso di sede di servizio ordinaria e da uno a due nel caso di sedi disagiate. Interveniamo con l'obiettivo di garantire che il personale in prima assegnazione possa contribuire a migliorare l'efficienza degli uffici ove presta servizio. Inoltre, per la Polizia di Stato è prevista una riduzione della durata dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di commissario, di vice commissario, di commissario tecnico, con una correlativa estensione in alcuni casi della durata del tirocinio. L'articolo 2 riguarda l'ordinamento e l'organizzazione dell'Arma dei carabinieri e interviene sulla disciplina e sull'organizzazione mobile e speciale dell'Arma, che sarà articolata nel comando unità mobile e nel comando unità specializzate. un assetto ordinativo introdotto nel 2022 per rendere più efficiente l'attività di comando e controllo. L'obiettivo è quello di riunire le funzioni per recuperare una posizione relativa all'incarico di *privacy* La rimodulazione delle due posizioni di vertice comando unità mobile e comando unità specializzate, che potranno essere istituite successivamente anche attraverso il loro accorpamento, porterà al recupero di una posizione di generale di corpo d'armata da destinare proprio all'incarico del *privacy* Come sappiamo, ai compiti istituzionali dell'Arma dei carabinieri quale forza militare di polizia si affiancano peculiari e importantissimi compiti nel settore della tutela ambientale e forestale: un insieme di attività e competenze che si traduce in un fondamentale e determinante contributo offerto dall'Arma, in linea con la finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, volto alla realizzazione della transizione ecologica, della neutralità climatica e dello sviluppo ambientale sostenibile. Grazie a questo provvedimento, su un conto corrente dedicato andranno le somme maturate a titolo di IVA a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione delle biodiversità, già affidate al Corpo forestale dello Stato. estesa inoltre, per un ulteriore triennio 2024-2026, la riduzione a trenta giorni dei periodi minimi di comando, di attribuzione delle specifiche di servizio e di imbarco validi ai fini dell'avanzamento. In questo modo viene garantito un adeguato margine di flessibilità nei casi di incarichi di comando o di attribuzioni specifiche riguardanti sopravvenute ed imprevedibili evenienze: una modifica necessaria per evitare che elevate professionalità, a seguito di impiego esterno rispetto all'amministrazione militare e dell'acquisizione di ulteriori competenze, optino per lasciare il servizio alle dipendenze dello Stato, così vanificando e disperdendo l'esperienza conseguita e maturata. Vengono chiariti i dubbi interpretativi relativi alle promozioni di tenenti colonnelli; l'articolo 5 punta al riordino e alla riorganizzazione anche sotto il profilo ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In materia di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene riconosciuta una quota dei compensi spettanti, che quindi non affluisce al fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato. Viene anche autorizzata l'assunzione, fino a 54 unità, per la qualifica iniziale del ruolo di ispettori antincendi mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso interno del 2023. L'articolo 6 potenzia, per un totale di 128 unità, il contingente extra-organico, il cosiddetto contingente speciale del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, al fine di rafforzarne l'attività in materia di prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Si interviene anche sul personale del Corpo delle capitanerie di porto e Guardia costiera, con il fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare. prevista così la possibilità di destinare quattro unità del personale fuori dal territorio nazionale per l'impiego presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari in qualità di esperti. In questo modo si potranno promuovere attività di supporto e consulenza su atti di amministrazione marittima. L'evoluzione tecnica della materia relativa alla sicurezza del trasporto marittimo, *safety* e *security* ambientale, nonché le complesse norme sull'imbarco e sbarco dei marittimi, prevedono la conoscenza di norme nazionali, europee e internazionali, richiedendo uno spinto approccio tecnico-amministrativo fondamentale per agevolare il proprio naviglio di bandiera ad effettuare operazioni commerciali rapide e veloci. Avremo l'indubbio beneficio sia di agevolare l'attività dei rappresentanti diplomatici, sia di velocizzare e snellire le pratiche amministrative, con evidenti ripercussioni positive sulla sicurezza dei traffici e sulla velocità delle operazioni commerciali. In materia di benefici assistenziali, è prevista la trasformazione del fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in una fondazione con compiti come l'assistenza agli orfani del personale, l'assistenza scolastica a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, contratti su assicurazioni, sovvenzioni per gravi malattie e onerosità delle cure. Infine, vogliamo istituire la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere, un obbligo morale da parte nostra, un indubbio riconoscimento per ricordare, con manifestazioni e cerimonie, chi con il suo sacrificio consolida l'identità nazionale. L'attenzione del Governo Meloni per il comparto è dunque concretamente dimostrata dalle ingenti risorse stanziate con il potenziamento degli organici attuati in precedenza. Con il provvedimento di carattere ordinamentale che ci apprestiamo a votare oggi dimostriamo una volta di più l'attenzione che stiamo dedicando all'intero settore di sicurezza e soccorso. Lo Stato è ogni giorno concretamente al fianco di chi quotidianamente difende e protegge i cittadini scelta che dovrebbe unire tutto il Parlamento per chi veste una divisa e rappresenta lo Stato.

e gli spunti che sono stati forniti dai rappresentanti delle rispettive Forze di polizia e Forze armate. In questo solco, ben venga un provvedimento che si occupi di dare risposte precise e di fornire finalmente una soluzione pratica alle storture o comunque alle disposizioni che nel tempo si sono rivelate non più rispondenti alle esigenze dei rispettivi Corpi. In questo senso, quindi, una esigenza di semplificazione, di razionalizzazione e anche di adeguamento delle norme si pone sicuramente nel solco di una ottima tecnica legislativa, di un intervento che, anche dal punto di vista politico, non può che essere favorevolmente accolto e valutato.

di riguardo nei confronti delle sedi disagiate, in maniera tale che si favorisca un ricambio, si invogli il personale a sceglierle, nella consapevolezza che potranno essere poi riassegnati più velocemente. Si accolgono anche con favore, le norme relative alla riduzione dei tempi per lo svolgimento dei concorsi per vice commissario e commissario, iscrivono nell'ottica della semplificazione. Allo stesso modo si accolgono favorevolmente anche le norme relative agli spostamenti che possono essere fatti in deroga alle regole ordinarie nella contingenza del Giubileo,

dei contributi economici in favore delle famiglie delle vittime del dovere, del terrorismo e delle organizzazioni criminali, perché è una norma che alla fine non avrebbe impegnato particolari risorse e sarebbe servito a dare una misura di attenzione specifica

le celebrazioni per la commemorazione delle vittime. Anche questa è una misura che lascia il senso delle cose un po' incompiute, soprattutto in considerazione degli scenari di guerra che ci attanagliano e in considerazione dell'impegno delle Forze armate, sempre maggiore nello scenario internazionale, e senza trascurare, né dimenticare che domani ricorre l'anniversario della strage di Nassiriya *(Applausi)*, dove persero la vita ben 17 militari e fra essi ricordo il maresciallo Alfio Ragazzi e il sottotenente Giovanni Cavallaro, originari entrambi di Messina. di Messina. Le famiglie di queste vittime, che subiscono la perdita dei loro cari, hanno diritto a che queste commemorazioni vengano fatte con una necessaria e doverosa dotazione economica, proprio perché non sia soltanto una celebrazione fine a se stessa. Su questo devo dire che si infrange la buona volontà del Governo, che alla fine adotta dei provvedimenti, ma sembra non essere mai in condizioni di dar loro quello spunto finale, che farebbe finalmente decidere anche questo Gruppo e questa parte di opposizione per un voto favorevole. Invece, siamo costretti ad un voto di astensione, considerato costruttiva nella parte in cui, comunque, c'è un riordino, una semplificazione e un adeguamento di misure, anche in considerazione delle necessità di organico che si profilano, dell'aumento della dotazione del contingente speciale dei carabinieri che si occupano della tutela del patrimonio culturale dello Stato e anche della parificazione del trattamento retributivo fra agenti donna e agenti di uomini della Polizia penitenziaria. Pensare di essere arrivati al 2024 per sancire che in una pubblica amministrazione uomini e donne debbano prendere gli stessi stipendi, è davvero il segnale che c'è un *gender gap* che va colmato quanto più velocemente però, ci sono altri aspetti, come appunto scarse misure economiche, poca attenzione nei confronti delle vittime del dovere e dei loro familiari, per i quali non ci sentiamo di esprimere un voto favorevole. È però un'astensione che vuole incoraggiare il Governo a essere più responsabile e a voler essere anche più coraggioso nelle misure che adotta; determinate strategie che, francamente, hanno il senso di una manovra populista. Continuare a portare gruppetti di migranti avanti e indietro dall'Albania, impegnando importanti risorse, e lasciare senza risorse, invece, provvedimenti che farebbero davvero la differenza, è il segnale che non c'è una politica reale. È una politica di cui siete voi soltanto interpreti, mentre l'opposizione vive in una torre eburnea. La gestione delle risorse non soltanto deve essere razionale, ma deve essere anche parametrata alle effettive necessità e al sentire effettivo delle Forze armate e dei loro appartenenti.

è un importante disegno di legge, che è ancora all'esame delle Commissioni 1ª e 2ª del Senato e che è stato approvato alla Camera, che riguarda una serie di interventi volti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, con l'inasprimento di pene e con un'estensione di misure che cercano di sanzionare in maniera più efficace comportamenti lesivi dell'ordine pubblico e con maggiore tutela del personale. Noi siamo, infatti, dalla parte del popolo in divisa. Vi è chi sabato, a Bologna - centri sociali ed estrema sinistra - ha ferito ancora una volta poliziotti e carabinieri e poi c'è chi per tutelarli. Quindi, quel disegno di legge è importante. Quest'altro disegno di legge, dedicato al comparto sicurezza-difesa, in estrema sintesi, prevede interventi riguardanti l'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Non dobbiamo mai dimenticare il soccorso pubblico per il contributo essenziale che dà nella vita ordinaria e, ahimè, anche straordinaria, rispetto alle calamità e agli eventi che colpiscono l'Italia. Ci sono nuove norme per dare tutela a chi tutela i cittadini. Abbiamo arricchito il testo, con emendamenti e con varie osservazioni. Per la Polizia di Stato si interviene sui tempi minimi di permanenza nella sede di prima assegnazione si rinnova un meccanismo che aveva dimostrato di essere poco efficace, per quanto riguarda l'assegnazione del personale di nuova nomina. sugli istituti superiori di polizia: sulla scuola superiore di polizia, che sarà diretta da un prefetto. Si interviene sul fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, che viene trasformato in una fondazione. Ci sono interventi che riguardano i carabinieri: gli assetti organizzativi del comando unità mobili, il reparto dei carabinieri in comando presso la Banca d'Italia. Vi sono altre assunzioni per la tutela del patrimonio culturale, 138 assunzioni di personale non militare: operai da utilizzare nell'Arma, visto che l'Arma ha assorbito il Corpo forestale dello Stato e, all'interno di quella struttura vi sono anche operai che devono provvedere a gestire alcune strutture in quell'ambito. Si agisce sulla Guardia di finanza, per quanto riguarda promozioni e sviluppo delle carriere; per il Corpo di polizia penitenziaria e, per quanto riguarda le Forze armate anche per i periodi di comando e i concorsi per i marescialli che abbiano una laurea o un'abilitazione professionale sanitaria. Come dicevo all'inizio, si interviene sul Corpo dei vigili del fuoco, sulle Capitanerie di porto e anche con la istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere. È un complesso, quindi, di norme. Questo provvedimento verte più sull'assetto organizzativo,

sono stati stanziati altri 100 milioni per gli straordinari delle Forze di polizia. Io stesso, insieme ad altri colleghi del Gruppo Forza Italia, ho presentato un emendamento per integrare con altri 30 milioni gli straordinari, perché ci sono le Forze armate che con Strade sicure e altre operazioni contribuiscono all'ordine pubblico e alla tutela dei cittadini. C'è quindi una massa di interventi tesi a rendere più certa la gestione dell'ordine pubblico,

anche misure organizzative per le nuove associazioni di stampo sindacale. È stata varata la legge, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale, ma, poiché bisogna rendere

vivere in maniera piena e rispettosa la nuova condizione di rappresentanza dopo la fase dei Cocer che ha ceduto il passo a questa nuova modalità. Si tratta, quindi, di un pacchetto di misure. Si può fare di più e di meglio, ma altri che oggi parlano non hanno rinnovato il contratto di lavoro. Ricordo che il contratto che noi rinnoviamo è quello che non hanno rinnovato quelli del Governo giallo-rosso, che evidentemente erano troppo attenti ai centri sociali e ad altre cose per pensare alle Forze di polizia. Noi, da quest'Aula, siamo solidali anche oggi con le Forze di polizia

non temiamo nulla, neanche il comizio della dottoressa Albano o il comizio di quell'altro di Bologna che ha preso la sentenza dalla sua conferenza di un anno fa con la frase sul nazismo e ha fatto copia e incolla. Forse dovrebbero fargli una trattenuta sullo stipendio. Ha riciclato qualcosa e dovrebbe avere 50 euro in meno.

Prisco e Perego quando ci sono state possibilità di confronto. Noi lavoriamo e andiamo avanti per il personale, per il popolo in divisa che anche io voglio ringraziare per la pazienza con cui sopporta le aggressioni e le centinaia di feriti. I provvedimenti che stiamo introducendo aumentano la tutela legale aumentano la tutela legale e sanitaria. Forse qualcuno sta dalla parte di chi ferisce le divise; noi stiamo dalla parte di quelle persone che hanno dedicato una vita allo Stato. Lo fece anche mio padre, che mi ha lasciato anni fa, e lo ha fatto anche mio fratello, con cui ancora condivido l'esperienza terrena. Lo ha fatto anche il padre della vice presidente Ronzulli, la quale prima ha dedicato a lui, che oggi compie

In Commissione, però, c'è stato un percorso abbastanza lungo e anche complesso che ha portato il provvedimento da cinque a diciannove articoli. Sono stati inseriti, grazie alla Commissione, numerosi nuovi articoli e numerose nuove disposizioni. Dichiaro fin da subito che il MoVimento 5 Stelle si asterrà su questo provvedimento, e il motivo è politicamente presto detto: non avete stanziato soldi, ce ne sono veramente pochissimi; non cambierete la storia delle Forze di polizia, di sicuro, e non renderete l'Italia un Paese più sicuro, al contrario di quanto è stato detto fino ad ora. Faccio un esempio: fate il gioco delle tre carte con lo spostamento di personale già presente per il Giubileo di Roma; il personale c'è già e lo spostate semplicemente a Roma. Ci sono poi disposizioni certamente meritorie, per l'amor del cielo, che riguardano il reclutamento dei congiunti del personale delle Forze di polizia e la loro partecipazione ai gruppi sportivi delle Fiamme Oro: sono familiari di vittime e quindi è giusto anche agevolarli con un percorso preferenziale nel reclutamento. Date però la possibilità agli psicologi presenti nelle Forze di polizia di poter esercitare anche in privato: non vedo come questo possa cambiare la sicurezza del Paese, ma tant'è, questo è quello che avete inserito. Si riducono i corsi di formazione del personale della Polizia di Stato, e immagino che anche questo lo riteniate utile. Avevo presentato un emendamento che chiedeva una verifica al 30 giugno 2025 per capire se tutte queste disposizioni che avete messo in atto siano o saranno funzionali, ma l'avete bocciato. Non so se avete già idea che non funzioneranno e quindi non vi serve verificarlo, oppure se siete così baldanzosi da sperare che questo cambi veramente le sorti della sicurezza del Paese. Io qualche dubbio Vengono disciplinate le promozioni: state disciplinando l'ovvio, visto che già mettete nero su bianco anche nella relazione il fatto che andate a sostituire i colonnelli con tenenti colonnelli, che già erano in vacanza. È come già state facendo ora: al 1° luglio di ogni anno c'è la verifica delle vacanze e quindi la promozione dei tenenti colonnelli. Ciò avviene già di fatto e semplicemente lo state riportando nero su bianco. Si permette ai Carabinieri di assumere personale operaio: è meritorio, ma anche questo credo che sarà ininfluente sulla sicurezza del Paese.

banalmente parametrato alle persone che usciranno dal servizio nell'anno precedente. Quindi assumete solo esclusivamente in numero inferiore o uguale al personale uscito dalla pianta organica. Avete inserito una delega per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Non potevate già farlo? Vi siete dati un'autodelega. Avevate Avevate inserito la trasformazione del Fondo di assistenza della Polizia di Stato, salvo poi votare contro quanto da voi stesso proposto. Quindi mi domando: avete sbagliato a proporlo o avete sbagliato a bocciarlo? *(Applausi)*. Non si capisce se siete nel pieno delle vostre facoltà, perché o l'uno o l'altro. brevemente anche sull'aumento della contribuzione obbligatoria per quel che attiene al Fondo di previdenza di Guardia della finanza, Polizia di Stato e Carabinieri:

che, per aiutare Guardia di finanza, Carabinieri e Polizia di Stato, questi debbono contribuire ulteriormente versando ulteriori fondi; cioè togliete dal loro stipendio per loro stessi. Credo che questa operazione non andasse fatta. O quantomeno se aveste ascoltato il consiglio di qualcuno dell'opposizione (il sottoscritto), avreste potuto almeno ascoltare le associazioni di categoria;

non erano neanche nostri (sto perorando la causa altrui, credendo che sia meritoria). Parlo delle misure in materia di stanziamenti per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti.

madre uccisi in servizio avesse la possibilità di ricevere un qualche aiuto, quantomeno per gli studi. Avete bocciato inoltre l'esenzione fiscale per quelle famiglie.

Concludo ringraziando anch'io le Forze di polizia e le forze del comparto difesa e sicurezza riportando le parole del senatore Gasparri. Anch'io dico loro grazie, ma grazie soprattutto perché riescono a sopportare tutti i santi giorni la propaganda che fate alle loro spalle. Dite di aiutarli, dite di essere al loro fianco, ma di fatto emanate questi provvedimenti che non servono a nulla. Per questo dichiaro ancora il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle.

oggi siamo chiamati a esprimere il nostro sostegno a un disegno di legge che segna un passo importante per il rafforzamento delle nostre strutture di sicurezza e difesa nazionale; un tema che ci sta profondamente a cuore e che rappresenta una delle colonne portanti della nostra azione politica. Questo provvedimento si pone l'obiettivo di rinnovare e potenziare l'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. il risultato di un lavoro attento e condiviso, nel quale il Gruppo della Lega ha svolto un ruolo determinante. Abbiamo lavorato in Commissione affinché il testo tenesse conto delle esigenze concrete di chi ogni giorno opera per garantire la sicurezza e la difesa del nostro Paese. Mi spiace della polemica che abbiamo sentito in Aula per la mancata approvazione di alcuni emendamenti. Credo che non possiamo non replicare ad una dichiarazione del collega Cataldi del MoVimento 5 Stelle riguardo alla maggiore sicurezza percepita dal cittadino se un ladro rimane un po' di più in carcere. Ebbene, questo quesito lo vorrei porre alla signora che la scorsa settimana, nella mia Provincia, è stata brutalmente malmenata nella sua abitazione, nonostante avesse indicato ai ladri dove teneva gioielli e denaro; di fatto se l'è vista davvero brutta. Difficilmente in quel caso i ladri sono persone spinte dal bisogno (è stato detto, infatti, che spesso sono persone spinte dal bisogno quelle che vanno a rubare nelle abitazioni).

dal fatto che nel momento in cui questi ladri, una volta catturati, vengano immediatamente rilasciati, se possa sentirsi rassicurata dal fatto che la giustizia interviene puntualmente per difendere i propri concittadini oppure se ritenga sia lassista con chi delinque. Ecco, io io penso che oggi cittadino meriti un'attenzione su quella che è la propria vita e meriti altresì che le pene abbiano il loro percorso proprio per garantire la sicurezza di tutti noi. Le modifiche introdotte con il provvedimento al nostro esame testimoniano l'impegno del nostro Gruppo volto a favorire un quadro normativo che sia all'altezza delle sfide attuali. In particolare il disegno di legge prevede interventi significativi per la struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri, razionalizzando la catena di comando per migliorare l'efficienza e ottimizzare le risorse con una gestione più puntuale nelle competenze. Allo stesso tempo viene affrontata la necessità di una maggiore protezione del nostro patrimonio culturale e naturale con l'istituzione di misure per la salvaguardia delle riserve naturali e dei beni culturali spesso esposti a minacce, con la necessità quindi di una tutela rafforzata. Il provvedimento dedica inoltre attenzione alle esigenze specifiche del personale in servizio, stabilendo condizioni più favorevoli per i trasferimenti, specialmente nelle aree più disagiate. Italia Viva direi che, ebbene sì, ci voleva proprio un Governo di destra per sancire la parità retributiva tra il personale maschile e quello femminile della Polizia penitenziaria modifiche contenute in questo disegno di legge che però, ahimè, vedrà l'astensione della sinistra in modo particolare, a quanto si è appreso, dei Gruppi MoVimento 5 Stelle e Italia Viva. Anche in questo contesto la propaganda rispetto alla parità di genere rimane con parole al vento, ma quando si tratta di approvare atti concreti vediamo che non si trasforma in voto. Ciò dimostra un impegno concreto per migliorare la qualità di vita dei nostri agenti e militari, contribuendo così ad una migliore stabilità e motivazione del personale. degli agenti aggiungerei anche quelle morali; ferite profonde che hanno tracciato un solco in una categoria che si sente poco tutelata in modo particolare da una certa parte politica, quella stessa parte politica riconducibile alla Salis, la stessa condannata per per resistenza a pubblico ufficiale; quella stessa parte politica che abbiamo visto manifestare contro le paventate norme liberticide che sarebbero state introdotte da questo Governo. parte politica che nei fatti vorrebbe impedire, attraverso i propri sindaci, l'autorizzazione a manifestazioni organizzate da chi non la pensa come loro. Ricordo bene la sceneggiata messa in campo dell'allora sindaco di Firenze Nardella sul convegno organizzato dalla Lega e sull'onda nera che avrebbe colpito Firenze. Ricordo il nostro pullman bloccato da un corteo non autorizzato. Tornando a quanto ci accingiamo a votare tra poco, questo disegno di legge rispecchia i valori che ci guidano e che ci spingono a lavorare instancabilmente per garantire sicurezza, efficienza e sostegno ai nostri corpi di difesa e sicurezza. Siamo convinti che queste misure contribuiranno a rendere il nostro sistema più moderno, più organizzato e meglio equipaggiato per affrontare le sfide del futuro. Per tutte queste ragioni annunciamo con convinzione il voto favorevole del Gruppo Lega, certi che il provvedimento al nostro esame rappresenti un ulteriore passo avanti per un'Italia più sicura e più forte. In ultimo, Presidente, per concludere, in merito ai fatti gravi di questi giorni, dove a Milano abbiamo visto un corteo inneggiare all'attacco antisemita di Amsterdam, quelli di Bologna, con il ferimento di alcuni agenti da parte degli antagonisti, a chi oggi continua ad agitare lo spauracchio dell'arrivo delle camicie nere, consiglio un buon oculista, visto che il colore delle camicie è rosso e direi di un rosso sangue simile a quello sui volti della presidente Meloni e del ministro Bernini apparso nei manifesti dei collettivi affissi a Bologna. Spero vivamente che il richiama alla rivolta sociale invocato da Landini non sia stato male interpretato. *(Applausi)*.

Signor Presidente, parto dall'ultima considerazione che ho ascoltato per dire che qui parliamo di questioni concrete che incidono sulla vita di professionisti

assistito in questi giorni a Bologna, cerchiamo di evitare lo scontro ideologico, concentriamoci sui temi concreti - come abbiamo fatto - e poi ci possiamo dividere e non essere d'accordo su una parte dei provvedimenti o su alcune norme che inseriamo. Ma lo scontro non serve ad aumentare le risorse per le Forze dell'ordine, che anzi rischiano di diminuire; non serve per costruire la cornice migliore per poterli far lavorare. parte del Gruppo Partito Democratico desidero rinnovare la fiducia alla Difesa italiana, alle sue donne e ai suoi uomini, alle nostre Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco. Non ci sia dubbio alcuno che il Parlamento - il Gruppo Partito Democratico in questo caso - è al loro fianco e non smetterà mai di lavorare per costruire le condizioni migliori anche nelle norme e nei provvedimenti per far sì che possano lavorare nella maniera migliore. È questo il faro che ci ha guidati nell'esprimere i nostri voti. Questo è un provvedimento che oggettivamente mescola tante cose diverse, anche un po' eccessivo; è una sorta di *omnibus* della sicurezza e della difesa, dove, se avessimo lavorato sui singoli temi in provvedimenti *ad hoc*, probabilmente avremmo fatto un miglior lavoro. Si mescolano questioni condivisibili con alcune esigenze molto parcellizzate e singole di alcuni gradi e di alcuni ruoli delle forze della della Difesa e molto spesso anche gli interventi più giusti mancano di coperture finanziarie, cioè non facciamo le nozze coi fichi secchi. Ci sono ambizioni che, però, non sono seguite da una copertura finanziaria, da risorse utili per mettere in grado le Forze dell'ordine, le forze della Difesa di poter fare

nel caso delle sedi disagiate), così anche come le deroghe parziali. Certamente bisognerà lavorare sul Giubileo per avere una maggiore flessibilità. Ma concordo con il collega

avuto incidenti sul posto di lavoro e quindi è giusto metterle in grado di avere criteri diversi di accesso, così come condividiamo la norma sugli psicologi. Altre norme funzionano solo a metà,

del Corpo forestale sotto i Carabinieri, costruendo un nucleo *ad hoc*, abbiamo aumentato le funzioni,

nelle foreste, nei boschi. È un lavoro enorme, radicato su tutto il territorio nazionale, che non ha però risorse a sufficienza per essere portato a termine. Questo vale anche per i beni culturali. Cosa non ci convince, dove manca un'attenzione sufficiente? Non ci convince il lavoro fatto un po' a spizzichi e bocconi sugli avanzamenti di carriera, su quando scattano le promozioni, perché scattano solo su alcuni gradi e non su altri; anche il lavoro fatto sui corsi di formazione non ci sembra sufficiente e avrebbe avuto bisogno di una maggiore riflessione. però, di due temi su cui avremmo costruito proprio una disciplina *ad hoc.* Sul Corpo della polizia penitenziaria quanti dibattiti abbiamo fatto in

tra uomini e donne all'interno della Polizia penitenziaria (quello era stato già fatto precedentemente): si è solo detto che si aumentano le possibilità dei profili femminili di lavorare dentro gli istituti penitenziari, chiarendo, con una norma evidentemente di buon senso e normale, che tutti comprendono, che nelle attività di monitoraggio e sorveglianza nelle unità detentive maschili e femminili ci lavora personale maschile e femminile.

Come dicevo prima, alcune misure, anche condivisibili, non hanno le risorse necessarie per poi funzionare. Sul tema dei Vigili del fuoco siamo d'accordo nell'aprire ad una nuova ad una nuova delega: è un tema necessario e da questo punto di vista c'è da fare una riflessione che spero si farà all'interno della delega. Con tutto il tema della transizione energetica e della lotta ai cambiamenti climatici e delle emergenze di protezione civile, capire come noi dotiamo di nuovi compiti, di nuove risorse e anche di personale necessario anche specializzato

penso che facciamo un'operazione parziale e anche un po' "pelosa". Io ho l'impressione che, quando facciamo questo, dobbiamo affiancarci degli strumenti concreti. Ed è assurdo che voi abbiate rifiutato di votare degli emendamenti semplici, con una minima copertura finanziaria, come quello da tre milioni di esenzione fiscale per aiutare e sostenere coloro che hanno perso un proprio caro nell'attività di servizio e un milione per borse di studio per i figli delle vittime del dovere. Su questo, oggettivamente avete perso un'occasione per dare un segnale importante sul fatto che il Giorno del ricordo delle vittime del dovere non è solo non è solo un'occasione retorica, ma è anche un'occasione concreta per ricordare chi si spende per noi.

riflettevo su un intervento che, per quanto politico, essendo fatto e promosso da questo Governo, era destinato a svilupparsi su ampi tratti tecnici ed economici, quando mi sono imbattuta nelle tragiche immagini che provenivano dalla piazza di Bologna e nella violenta aggressione subita dai nostri ragazzi in divisa. A questo punto mi obbligo a non tacere su questi fatti: non accettiamo e non accetteremo più le giustificazioni agli aggressori con la solita litania che si è trattato di una risposta politica a un corteo di provocatori. Vogliamo liberarci dal farisaico rispetto a senso unico delle idee degli altri e chiamare le cose con il loro nome. Credo che sia l'ora di definire i personaggi che si sono resi protagonisti dell'aggressione con il loro nome, cognome e aggettivo qualificativo. I soggetti che hanno vigliaccamente aggredito le Forze di polizia si devono definire delinquenti, senza se e senza ma. *(Applausi)*; una violenza brutale, una caccia all'uomo in divisa, ostaggi di un odio che va etichettato così come appare, anche se la cosa dà fastidio, perché c'è chi si contraddice. Tanta ipocrisia, tante illusioni, tanta comodità. Ma non possiamo cedere e considerare la "contromanifestazione" - come viene chiamata dalle forze che si autoproclamano democratiche in quest'Aula - un diritto ad esserci in quella piazza, perché non vi è diritto e mai ci sarà - a colpire le Forze dell'ordine che quotidianamente garantiscono - mi ripeto - l'ordine sociale; quell'ordine che i cosiddetti democratici ripudiano; quell'ordine che chiedono di osservare solo quando a comandarlo sono loro. Giustificare o, peggio ancora, tacere sugli incresciosi fatti significa esserne complici. La più attenta cifra di questa complicità sta proprio nel continuare a tacere sui gesti di quei facinorosi e alimentarne le gesta, con la solita scusa che è stata la legittima reazione al fascismo dilagante, l'invio delle 300 camicie nere e tante altre cose che abbiamo letto nelle agenzie in questi giorni. Nello Stato democratico in cui crediamo

di frapporsi legittimamente a una violenza che viene artatamente e spudoratamente nascosta sotto l'egida di un'ideologia. Qui si genera il cortocircuito: scendono in piazza con le magliette di Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa, le gonne arcobaleno, magari *made in China* e fabbricate dai ragazzini pagati a poche monete, con il solo manifesto intento di picchiare selvaggiamente chi si frappone legittimamente alla loro guerriglia e a chi cerca di tutelare non solo il diritto di tutti a manifestare manifestare le proprie idee, ma anche il diritto di pari rango dei cittadini di Bologna, avulsi completamente da quell'agone, di camminare liberamente per la loro città, forse anche semplicemente per quelle famose boccate d'aria che in tanti periodi non erano possibili. Il silenzio glaciale delle istituzioni di quella città non ci sorprende. A dire il vero, in taluni casi il silenzio sarebbe stato oro, perché certe frasi scombinate del primo cittadino possono essere clinicamente osservate e studiate; o la partecipazione in quel contesto della segretaria del Partito Democratico, che ribadisce il silenzio glaciale e che non sorprende questa parte dell'Aula. Del resto, il venerdì precedente, un altro alto esponente di quelli che si ostinano a chiamarsi democratici aveva incitato un'altra piazza, *apertis verbis*, alla rivolta sociale, a scardinare lo Stato con atti di violenza - perché la rivolta non è mai pacifica - per affermare le proprie idee, a sciogliere il patto sociale, a distruggere il Leviatano, a dare il via libera al detto di Plauto ripreso da Hobbes che ogni uomo è un lupo per un altro uomo. Anche in questo caso, nessuno dei sodali a quel Masaniello ha gridato allo schifo o allo scandalo; ma anzi, anche in quel caso, le sconsiderate affermazioni sono state oggetto di rivendicazione da parte dell'autore e di giustificazione da parte del partito che lo esprime, ma giustificato incondizionatamente. La magistratura, di cui abbiamo sufficientemente parlato, che in questi casi ha l'obbligo di aprire un fascicolo, saprà sopire quelli che auspichiamo siano contenuti nell'alveo di un delirio. Ma oggi, per il qui ed ora, oltre a ribadire il nostro biasimo per i fatti di Bologna, vogliamo testimoniare il nostro impegno per le Forze dell'ordine, per l'Esercito, per i Vigili del fuoco e lo facciamo con questo provvedimento, in cui inseriamo, ad esempio, considerata la complessità del ruolo che quelle persone ricoprono, all'articolo 11, il riconoscimento economico e il 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture per il personale che svolge funzioni tecniche nell'ambito delle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, adeguandosi a quanto prevedono gli allegati I.10 del codice degli appalti inoltre inserito le assunzioni per il personale del Comando dei carabinieri, sia per quanto previsto dall'articolo 6, per il Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e artistico, dove la norma in esame incrementa di 8 unità i tenenti colonnelli, 22 gli ispettori, 5 sovrintendenti e 10 carabinieri appuntati, sia per quanto inserito nell'articolo 10, che prevede finalmente l'assunzione di un massimo di 100 unità per l'anno 2025 e di 38 per l'anno 2026 di personale operaio a tempo indeterminato. In In aggiunta ricordo le disposizioni fondamentali previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale si autorizza l'assunzione fino a 54 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, scorrendo la graduatoria di concorso interno del 2023. Si affronta la sicurezza del prossimo Giubileo, per il quale si deroga in materia di permanenza e trasferimenti. Si determinano i criteri di istruzione, ma soprattutto, con l'articolo 12, si delega il Governo ad emanare entro un anno la determinazione di disposizioni integrative e correttive concernente le funzioni e l'ordinamento del Corpo. Vado a concludere, Presidente, ma non posso tralasciare le importanti modifiche riguardanti diversi fondi di assistenza, cassa e fondo previdenza, enti e circoli Per taluni non è abbastanza o forse dall'attico newyorkese non vedono cosa avviene nella realtà. Per altri, questi articoli sono stati presi come numeri su una pagina bianca scritta dalla politica. Queste parole, però, sono importanti non solo per gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine, dell'Esercito, dei Vigili del fuoco, ma anche per le loro famiglie, per quei figli inconsapevoli mentre frequentano l'asilo, aspettano con un orsetto con la divisa della nostra Patria il ritorno della madre dalle missioni. Sono importanti per quelle donne, quelle ragazze che, seppur orgogliosamente consapevoli dell'uomo che hanno scelto, si trovano a fare la prima ecografia per il primo figlio da sole, perché quell'uomo magari è impegnato in qualche piazza a prendere delle vigliacche sassate. Ai propri uomini e alle proprie donne questo Governo sta vicino non solo con le parole, ma soprattutto con i fatti, i fatti contenuti È per questo motivo, per tutti questi motivi, che orgogliosamente esprimo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

vorrei richiamare l'attenzione su quello che è avvenuto oggi a Milano, dove, al *murale* dedicato alla senatrice a vita Liliana Segre e a quello di Sami Modiano è stato fatto uno sfregio enorme. È l'ennesimo atto di antisemitismo dopo i fatti gravissimi che ci sono stati ad Amsterdam, che tutte le forze politiche hanno condannato; un antisemitismo che è dilagante, spaventoso, che ci vede tutti impegnati. Su questo credo che tutti dovremmo essere uniti in un'unica battaglia. Fatemi, però, ringraziare le Forze dell'ordine, perché in molte manifestazioni dove si scende in piazza con la bandiera della pace, spesso e volentieri, invece di inneggiare alla pace, si inneggia all'odio, si inneggia alla caccia, si inneggia contro chi è diverso. Invio un abbraccio, da tutto il nostro Gruppo, ma voglio immaginare e ben credo di tutta l'Aula, alla senatrice Segre e a Sami Modiano, che con coraggio, tutti i giorni, continuano a raccontare quello che i loro occhi sono stati costretti a vedere.

Presidente, intervengo su un argomento importante, riguardante l'amministrazione della giustizia, che è la manifestazione indetta dall'ordine degli avvocati di Roma, di tutto il Lazio e non solo, anche di Torino,

il dibattito che si è tenuto in quest'Aula, sulla questione della magistratura e non solo, mi obbliga a intervenire per dire: cari colleghi della maggioranza, fermatevi. maggioranza, fermatevi. I toni che sono stati usati in quest'Aula sono assolutamente inaccettabili. Vi richiamate spesso alle democrazie occidentali, ma siete fuori dalle democrazie occidentali. Sono democrazie liberali, dove c'è la separazione dei poteri, finora.

sono inaccettabili. *(Applausi)*. Tra l'altro, ai maestri improvvisati del garantismo vorrei ricordare che il principio su cui si appunta il garantismo, la difesa di tutti quelli che devono essere garantiti, è il rispetto della legge, non il rispetto delle maggioranze; non è il rispetto di chi ha il potere, anche se ottenuto con il voto. Questo è il garantismo. E non possiamo sentire i toni usati nei confronti del sindaco di Bologna, definito caso psichiatrico. psichiatrico. La delegittimazione dell'avversario politico con questo tipo di attacco è foriera di qualcosa che non vorremmo né vedere né sentire. definire uno dei principali esponenti del sindacato italiano, Maurizio Landini, un Masaniello, quando ancora ricordiamo l'attacco alla sede della CGIL, quando ancora ricordiamo l'attacco alla sede della CGIL, rispetto al quale è stata inflitta qualche condanna, non soltanto giudiziaria, oltre che per gravi reati, anche da parte di tutti noi. Colleghi, davvero io vi invito tutti a una riflessione, perché i toni della discussione che c'è stata oggi non sono accettabili. Non sono quel presupposto indispensabile per la democrazia di questo Paese e per la dignità di questo Parlamento. Se, invece, qualcuno vuole sostenere che c'è un altro modello di Stato che si intende perseguire, ma anche praticare, da quello che vediamo in quest'Aula, lo dica con estrema chiarezza. Ma, con altrettanta chiarezza, noi, da questo punto di vista, siamo fermamente all'opposizione.

mi ero prefissato affinché resti agli atti. Sono molto sconcertato da quello che sta accadendo. Abbiamo assistito a una serie di sentenze similari, alcune con contenuti tratti da relazioni scritte da questi magistrati in precedenza. Mi riferisco a quella di Bologna, con riferimento alla Germania nazista, che era simile a quella che lo stesso magistrato aveva utilizzato in una conferenza un anno prima. Ciò fa immaginare che siano tesi

La dottoressa Albano ha attaccato pubblicamente il Presidente del Consiglio dicendo addirittura che alimenta violenza o altre cose. Siamo quindi al ribaltamento della realtà. Ho letto sui giornali frasi molto allarmanti di questa persona, che ieri ha anticipato la sentenza di oggi dicendo che un giudice monocratico aveva depositato un verbale e facendo trasparire l'esito. Ho chiesto, e lo ribadisco in Aula, un'ispezione per capire come funziona. Si consultano, si passano le carte, c'è un archivio comune? Non lo so, non faccio il magistrato e non ho idea di come funzionino le cose. Ho visto il caso Striano partire dalla procura nazionale antimafia e ho visto tutte le varie intercettazioni. Ho visto tante cose. Vorrei che ci fosse un po' di chiarezza sui comportamenti del giudice Albano, del giudice di Bologna e di altri, come quello che mandava le *mail* alla sua *mailing list* di Magistratura democratica,

in conflitto con i principi di uno Stato democratico, costituzionale e liberale. Mi auguro che la ripartizione dei poteri, che da Montesquieu ad oggi dovrebbe vigere tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario, possa essere ripristinata in questo Paese. Questa divisione tra poteri è messa a dura prova a Bari, così come a Bologna, a Roma e altrove. Sono esterrefatto, perché l'uso politico della giustizia continua e si manifesta giorno dopo giorno. Vorrei che tutti i colleghi si unissero alla nostra preoccupazione e all'invocazione di una riforma perché, al di là della separazione delle carriere, serve una rifondazione seria della magistratura. Abbiamo visto in questa legislatura, anche in Commissione antimafia e altrove, atteggiamenti di astio di persone che prima disponevano della libertà delle persone e che oggi vorrebbero indagare sul loro passato passato nel ruolo di parlamentari e che, quando si parlano tra di loro, danno dei giudizi sprezzanti anche su componenti di questa Assemblea. La storia è lunga e ne vedremo delle belle. Ne ho già viste delle belle, ma quelle che vedremo saranno ancora più belle.